in sede di esame del disegno di legge n. 1756 «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 6 dicembre 2006»;

Signor Presidente, il disegno di legge in titolo concerne l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra Italia e Moldova sulla cooperazione nel campo della difesa, sottoscritto a Roma nel 2006. Una iniziativa legislativa era già stata presentata dal Governo nel corso della passata legislatura e non ha potuto terminare l'*iter* a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere. delle Camere. Nel preambolo, l'intesa ribadisce l'adesione ai princìpi dettati dalla Carta delle Nazioni Unite e dall'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e cooperazione in Europa, adottato a Helsinki nel 1975, in un'ottica di sviluppo della cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate, onde consolidare le rispettive capacità difensive e contribuire al raggiungimento dello scopo comune di rafforzare la sicurezza e la stabilità in Europa.

Come sicuramente i colleghi senatori sapranno, esiste una parte del territorio moldavo che non è sotto la giurisdizione del Governo centrale di Chisinau: sto parlando della Transnistria. ha a che fare con gli armamenti e individua anche ambiti e forme di cooperazione tra i due Paesi, tra cui sicurezza e politica di difesa, *peace keeping* e operazioni umanitarie, abbiamo ritenuto opportuno ribadire che esiste il problema della Transnistria, una parte del territorio che si è proclamata indipendente nel 1990 e che da allora non ha mai consentito ad altri che al proprio "Governo"

congelati, che da quel lembo di terra che costeggia il fiume Nistro passano armi, droga, esseri umani e qualsiasi merce, in entrata e in uscita, che poi ritroviamo sui mercati, non soltanto europei ma, se penso alle armi, molto spesso dell'Asia centrale e anche dell'Africa. Quindi, quel che noi abbiamo voluto in qualche modo significare con questo ordine del giorno è la necessità di ricordare che esiste un problema in quella parte del mondo e che è in corso dal 2005 un negoziato nel formato cosiddetto 5+2, tra Russia, Ucraina, Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), Moldova, Transnistria, più Stati Uniti ed Unione europea che fungono da osservatori, che ha appunto come oggetto il futuro *status* della Regione. La situazione della Transnistria è seguita attentamente dall'OSCE, che opera in Moldova dal 1993 con la finalità di creare le basi di un dialogo politico e favorire i colloqui tra le parti, oltre che fornire assistenza tecnica e finanziaria per la distruzione degli armamenti, eredità dell'Unione sovietica. Una risoluzione pacifica e concordata del conflitto in Transnistria rappresenta un interesse strategico per l'Unione europea, anche in un'ottica di tutela della stabilità del vicinato europeo e di prevenzione dei rischi legati al crimine organizzato in materia di armi e contrabbando. Attualmente, tra l'altro, è presente in Transnistria un contingente militare russo in missione di pace, che è a presidio dei depositi militari ereditati dall'URSS. La richiesta di questo ordine del giorno nei confronti del Governo è di adoperarsi affinché nelle opportune sedi internazionali, e segnatamente mediante l'essenziale ruolo dell'OSCE, venga affrontata la questione del conflitto tra la Repubblica di Moldova e la Transnistria, al fine della ripresa di un negoziato stabile e di intraprendere, nell'attuazione dell'Accordo, tutte le iniziative atte ad impedire che materiali di armamento possano essere utilizzati in tale Regione. Come voi sapete, si sono tenute da poco le elezioni politiche in Moldavia. Vi è stato il passaggio di testimone da quello che potremmo chiamare un centrosinistra, ma che insomma era l'eredità del vecchio partito comunista, a un Governo di tipo diverso, che magari è più attento a questioni relative a ciò che l'Unione europea da sempre rappresenta, e cioè il rispetto delle norme internazionali, e quindi vi potrebbero essere le condizioni politiche generali per poter finalmente dare un impulso maggiore a questo tipo di trattati. Riteniamo che il Governo italiano, da sempre vicino alla risoluzione pacifica dei conflitti e anche interessato a ciò che avviene sul Mar Nero, dove appunto la Transnistria si affaccia tra la Moldavia e l'Ucraina, possa giocare questo ruolo all'interno dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa. Auspichiamo quindi che l'ordine del giorno venga giudicato accoglibile.

sottolineando come l'Italia segua la situazione in Transnistria; in particolare noi auspichiamo che i negoziati possano riprendere nel formato 5+2, con un ruolo rafforzato dell'OSCE. L'Organizzazione può infatti vantare, grazie ad una significativa presenza sul territorio che risale al 1993, una conoscenza della problematica superiore a qualsiasi altra organizzazione internazionale. quindi, guarda con favore alle mediazioni fin qui svolte, anche grazie al ruolo e all'impulso recentemente avuto da Mosca, e ci auguriamo che in un prossimo futuro risultati concreti risultati concreti possano essere riportati in una cornice che veda una maggiore responsabilità e presenza dell'OSCE sul territorio.

alla ratifica dell'Accordo. Accogliamo innanzitutto con favore il riferimento contenuto nel preambolo ai principi dettati dalla Carta delle Nazioni Unite e dall'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e cooperazione in Europa del 1975, poiché tale adesione chiarisce come la cooperazione fra le Forze armate sia esclusivamente volta al mantenimento della pace nella nostra Europa, che non è quella che si esaurisce con i confini dell'Unione europea, ma che comprende geograficamente e culturalmente anche i Paesi non membri dell'Unione europea come la Moldova. Il carattere non aggressivo dell'intesa è sottolineato inoltre dagli articoli successivi all'Accordo, che individuano nel *peace keeping* e nelle operazioni umanitarie le uniche fattispecie concrete di missioni che possono essere svolte congiuntamente dalle nostre Forze armate e da quelle moldave. A tale proposito, non posso che rilevare ancora volta, cari colleghi, come, mentre continuiamo a ribadire la nostra adesione ad accordi che hanno ad oggetto solo ed esclusivamente missioni di pace - ripeto: di pace - nella pratica poi partecipiamo a missioni il cui carattere pacifico non pare poi così lampante. Mi riferisco, ovviamente, cari colleghi, all'Afghanistan, dove la nostra presenza pare più inserita in un contesto di guerra che in uno di pace. Sono mesi che lo denunciamo. Abbiamo avuto il coraggio di presentare un ordine del giorno bocciato da tutte

davanti al ministro La Russa. Sono mesi che denunciamo questa circostanza del contesto di guerra e non di pace denunciamo che ogni tragico evento - negli ultimi giorni hanno assunto una cadenza quasi settimanale - ci fa sentire come Cassandre impotenti di fronte all'ostinata miopia di questo Governo e - lo ripeto - non solo

porremo al ministro La Russa. Tornando all'Accordo che ci apprestiamo a ratificare, vorrei soltanto sottolineare che esso non comporta oneri particolarmente pesanti per il nostro Paese, in quanto la stima prevista nel disegno di legge di ratifica è di 7.600 euro

rappresentante del Governo, colleghi senatori, il disegno di legge in esame reca l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata dalla Conferenza generale UNESCO il 2 novembre 2001. Tale Convenzione si è resa necessaria per ribadire l'importanza del patrimonio culturale subacqueo in quanto elemento importante della storia dei popoli e delle Nazioni. È convinzione condivisa che la collettività abbia diritto di beneficiare dei vantaggi educativi e ricreativi di un accesso responsabile e rispettoso del patrimonio subacqueo *in situ*. Vi è la consapevolezza che interventi non autorizzati sul patrimonio culturale subacqueo possano costituire una minaccia per quest'ultimo e nel contempo ne favoriscano il crescente ed inopportuno sfruttamento commerciale. Si ritiene che la cooperazione fra gli Stati, le organizzazioni internazionali, le istituzioni scientifiche, gli archeologi, i sommozzatori, le altre parti interessate ed il pubblico in generale, sia indispensabile per la protezione del patrimonio storico e culturale subacqueo. La Convenzione è uno strumento internazionale in grado di garantire la tutela dei beni culturali sommersi al di fuori della possibile zona di giurisdizione archeologica degli Stati costieri, colmando così le lacune ereditate dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982 e ratificata dall'Italia nel 1994. La Convenzione rappresenta un ragionevole compromesso tra le posizioni degli Stati, come l'Italia, che avrebbero voluto un'incondizionata estensione dei diritti dello Stato costiero sul patrimonio culturale situato sulla piattaforma continentale e nella zona economica esclusiva, e quelle degli Stati, tra i quali gli Stati Uniti d'America, che non erano disposti ad accettare la proposta indicata. Infine, si ricorda che la Convenzione in oggetto è entrata in vigore il 2 gennaio 2009. Entrando nel merito della Convenzione, essa definisce e delimita il concetto di patrimonio culturale subacqueo, includendo siti, strutture, edifici, resti umani, navi affondate ed il loro carico, oggetti preistorici. Con altrettanta chiarezza esclude dal concetto di patrimonio culturale subacqueo gli oleodotti, i cavi posizionati sui fondali marini ed altri impianti. La Convenzione definisce l'obbligo per le Parti di preservare il patrimonio culturale subacqueo nell'interesse dell'umanità e di adottare misure conseguenti e coerenti all'obbligo; indica prioritaria la conservazione *in situ* del patrimonio culturale prima di autorizzare o di intraprendere qualsiasi intervento su di esso; vieta lo sfruttamento a fini commerciali dello stesso; prevede un'attenta vigilanza degli Stati membri sul rispetto dei resti umani sommersi. mette in evidenza gli aspetti integrativi della Convenzione stessa rispetto alla citata Convenzione delle Nazioni Unite UNCLOS, precisando che le Parti possono autorizzare interventi sul patrimonio culturale subacqueo nella loro zona contigua, che non può estendersi oltre le 24 miglia marine dalla linea di base da cui si misura la larghezza del mare territoriale. Non vengono quindi pregiudicati i diritti, la giurisdizione e i doveri derivanti

non applicabili ad alcuna attività relativa al recupero di beni culturali, salvo che non vi sia una specifica autorizzazione da parte delle autorità competenti. Definisce la possibilità per gli Stati parte di stipulare accordi bilaterali, regionali e multilaterali e di sviluppare quelli già esistenti e norma il diritto esclusivo del singolo Stato a regolare il patrimonio culturale sommerso nelle acque interne, degli arcipelaghi e del mare territoriale. La Convenzione indica inoltre che la gestione e la tutela del patrimonio culturale subacqueo che giace nella zona economica esclusiva e sulla piattaforma continentale sono di pertinenza degli Stati cui pertengono cui pertengono le aree e sancisce che la tutela del patrimonio culturale subacqueo nell'area internazionale è in carico a tutti gli Stati parte, anche conformemente a quanto disposto dall'articolo 149 della Convenzione ONU sul diritto del mare. altresì le attività di cooperazione internazionale nelle operazioni di protezione del patrimonio culturale subacqueo, con riguardo ai settori dello studio, della ricerca e della conservazione, nonché dell'attività divulgativa; inoltre indicazioni circa la formazione in archeologia subacquea e le tecniche di conservazione del patrimonio culturale. Essa, infine, prevede l'istituzione o il rafforzamento di autorità nazionali competenti per la protezione del patrimonio culturale, che saranno responsabili della sua inventariazione, dell'effettiva protezione, della conservazione e della sua valorizzazione. Il disegno di legge n. 1739 chiede l'autorizzazione alla ratifica di questa Convenzione. L'articolato del disegno L'articolato del disegno di legge prevede che i compiti di tutela, inventariazione, conservazione e gestione del patrimonio culturale subacqueo siano affidati al Ministero per i beni e le attività culturali e che, per le navi di Stato o da guerra, le operazioni siano condotte in cooperazione con il Ministero della difesa. riferimento all'allegato alla Convenzione, che contiene 36 regole costituite da disposizioni pratiche molto dettagliate riguardanti le attività dirette alla tutela del patrimonio culturale subacqueo. Tali regole, largamente riconosciute ed applicate, sono diventate un punto di riferimento nel campo degli scavi e dell'archeologia subacquea e il loro inserimento nella Convenzione e nella ratifica viene ritenuto una fondamentale acquisizione. Il disegno di legge prevede inoltre il caso in cui la zona compresa tra le 12 e le 24 miglia nautiche si sovrapponga con analoga zona di un altro Stato con il quale non sia ancora attivo un accordo di delimitazione e dispone che gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa 12 miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale (la cosiddetta zona contigua) siano tutelati ai sensi delle «regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo», allegate alla Convenzione e già recepite dall'articolo 94 del decreto-legge 22 gennaio 2004, definisce poi la disciplina dei ritrovamenti nelle zone di protezione ecologica e contiene norme dettagliate riguardanti le denunce di ritrovamento e le richieste di autorizzazione. In particolare, esso ribadisce che i ritrovamenti effettuati nelle zone di protezione ecologica o sulla piattaforma continentale italiane devono essere dichiarati all'Autorità marittima entro 3 giorni e che l'autorizzazione all'intervento deve essere invece rilasciata, o negata, dal Ministero dei beni e delle attività culturali, cui vanno indirizzate le denunce e le richieste da parte dell'Autorità marittima. Si ritiene opportuno che anche il Ministero degli affari esteri debba esserne informato. inoltre che i ritrovamenti nell'area internazionale dei fondi marini e nel relativo sottosuolo o l'impegno a procedere ad interventi su tale patrimonio debbano essere denunciati al Ministero degli affari esteri, che è tenuto a trasmettere la denuncia al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché al Ministero della difesa se il bene in questione è una o da guerra. Esso indica infine nel Ministero per i beni e le attività culturali l'autorità competente per le operazioni di inventariazione, protezione, conservazione e gestione del patrimonio culturale subacqueo. La Relazione tecnica allegata al disegno di legge in esame, tenuto conto che la Conferenza degli Stati parte si riunirà almeno una volta ogni due anni a Parigi presso la sede dell'UNESCO, identifica quali oneri 6.330 euro per ogni biennio; nell'ipotesi che anche il Consiglio tecnico si riunisca in concomitanza con la Conferenza delle Parti, identifica 7.125 euro di oneri, sempre biennali. Il provvedimento è corredato da un'analisi dell'impatto della regolamentazione e di un'analisi tecnico-normativa, che forniscono un'ampia e dettagliata analisi del quadro normativo nel quale il provvedimento si inserisce, senza evidenziare problemi di incompatibilità.

la Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo è lo strumento internazionale per garantire la tutela dei beni culturali sommersi al di fuori della possibile zona di giurisdizione archeologica degli Stati costieri. Lo scopo è quello di migliorare il regime del diritto internazionale del mare, con riferimento alla protezione dei beni culturali. La Convenzione vincola e obbliga le Parti a preservare il patrimonio culturale subacqueo nell'interesse dell'umanità e ne vieta lo sfruttamento a fini commerciali; inoltre, sono gli Stati membri ad operare la vigilanza. La Convenzione incentiva la ricerca in questo settore e soprattutto la formazione di personale con competenze specifiche e metodologie atte alla conservazione dei siti. Qualificante è poi la costituzione negli Stati di autorità nazionali competenti per la conservazione, la protezione e la valorizzazione di tale patrimonio. Da parte del Gruppo della Lega Nord sarà quindi espresso voto favorevole, con particolare soddisfazione per l'aspetto che attiene alle sanzioni e quindi alla maggiore severità nei confronti di chi non rispetta il nostro grande patrimonio culturale subacqueo.